tenutasi il 22 e 23 ottobre di quest’anno nel collegio uninominale della Regione Lombardia n. 6, al fine dell’attribuzione del seggio resosi vacante per effetto del decesso del compianto senatore Silvio Berlusconi, sia presente - senatore della Repubblica il candidato Adriano Galliani. Al nostro nuovo collega formulo, a nome di tutta l’Assemblea,

Regolamento, sul disegno di legge n. 926 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 20242026». Invito il senatore Segretario a darne lettura.

bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni: per quanto attiene alla verifica di cui all’articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che il bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009. Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l’obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l’indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2023. In definitiva, si segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 199 miliardi per il 2024, dovuto a entrate finali pari a 688 miliardi e spese finali pari a 886 miliardi. Nel 2025 il saldo netto da finanziare è pari a 165 miliardi per effetto di entrate finali per 697 miliardi e spese finali pari a 862 miliardi. Nel 2026 il saldo netto da finanziare è pari a 132 miliardi con le entrate finali che si attestano a 711 miliardi e spese finali a 843 miliardi. Passando ai corrispondenti valori dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che nel 2024 le entrate finali per la pubblica amministrazione sono pari a 990 miliardi, le spese finali ammontano a 2023 miliardi e l’indebitamento netto si attesta su 92 miliardi; nel 2025 le entrate finali sono pari 1.042 miliardi, le spese finali ammontano a 1.123 miliardi e l’indebitamento si attesta su 80 miliardi; nel 2026 le entrate finali sono pari a 1.062 miliardi, le spese finali ammontano a 1.129 miliardi e l’indebitamento si attesta su 67 miliardi. Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall’articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l’indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2023, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2024. Si propone pertanto di sottoporre all’attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all’articolo 126, comma 4, del Regolamento.

pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell’ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell’esame parlamentare. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all’articolo 3, del Regolamento del Senato, si segnalano le seguenti disposizioni: - l’articolo 13, che al fine di agevolare la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni interviene apportando modifiche ad alcuni articoli del codice civile; - l’articolo 22, che interviene nel decreto legislativo n. 231 del 2007 (in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose) istituendo una banca dati informatica presso gli organismi di autoregolamentazione diretta a rafforzare il sistema di prevenzione del riciclaggio; l’articolo 72, comma 24, che individua quale centrale unica di committenza anche la “Centrale di committenza e stazione unica appaltante sisma 2016”, istituita presso la struttura commissariale ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n.189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari. Non si rinvengono, invece, nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale. Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione.

di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatta eccezione per le disposizioni segnalate nel predetto parere. Dispongo peraltro lo stralcio

(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) alla 5[a] Commissione, in sede referente, con il parere

dovranno comunicare i propri rapporti alla 5[a] Commissione entro venerdì 10 novembre. Le Commissioni sono sin d’ora autorizzate a convocarsi o ad integrare i propri ordini

che ipotizza un vero e proprio ribaltamento del rapporto tra Parlamento e Governo. Si tratterrebbe di una riforma, insomma, che vorrebbe passare dalla primazia del Parlamento e del pluralismo alla primazia del Governo e dell’uno. Signor Presidente, mi rivolgo a lei per rivolgermi ai colleghi senatori, perché a noi risulta che sia un annuncio e non sia ancora una riforma entrata in vigore e che

che noi ci auguriamo non veda mai la luce, ma è innanzitutto una mortificazione delle prerogative del Parlamento nonché dei diritti e dei doveri dei senatori. I senatori, infatti, quando esercitano le prerogative che la Costituzione riserva loro, non esercitano solo e tanto dei diritti che la Costituzione

Noi siamo molto preoccupati per la piega che sta prendendo la nostra democrazia parlamentare (Applausi), perché da un anno noi siamo chiamati solo a convertire decreti-legge.

che non si aggirino le norme regolamentari attraverso il collegamento di disegni di legge…

che dovrebbero escludere che vengano collegate alla legge di bilancio proposte di legge che, per esplicita previsione, non incidono sul bilancio, perché sono a invarianza di spesa. Fare questi collegamenti comporta che disegni di legge, come ad esempio quello sull’autonomia differenziata, che - ripeto - per esplicita previsione non comportano nessun incremento di spesa, vengano trattati durante la sessione di bilancio, sottraendo ulteriore tempo a un approfondimento, invece, doveroso. Questo spetta a lei, signor Presidente: garantire che le norme regolamentari vengano rispettate e che il collegamento con la legge di bilancio non venga costruito in maniera,

solo assicurarle che da parte della Presidenza del Senato vi sarà la puntuale osservanza di tutte le norme regolamentari. Mi permetto di segnalarle, perché siamo in una seduta ufficiale, che neanche è ipotizzabile che vi sia un divieto di presentare emendamenti e non mi pare, per la verità, che sia stato neanche lontanamente ipotizzato per quanto attiene le forze di opposizione. Le forze di maggioranza saranno in grado di valutare autonomamente e se vorranno presentare emendamenti, li potranno presentare.

Signor Presidente, essendo entrati nella sessione di bilancio ai sensi della comunicazione che ci è stata testé comunicata, non possiamo non evidenziare, intanto perché rimanga agli atti di questo ramo del Parlamento e poi affinché si possa anche aprire una discussione tra le forze politiche

di dover assistere ad un comunicato ufficiale del Governo nel quale, nell’annunciare l’invio del disegno di legge di bilancio al Parlamento, annunciava contemporaneamente la volontà di non presentare emendamenti da parte dei colleghi parlamentari di maggioranza. Nella fattispecie, evidentemente, il Presidente del Consiglio si è mosso contemporaneamente nella veste di Primo Ministro e di capo

un indirizzo di natura politica non può in alcun modo tradursi in una determinazione di natura giuridica. Ritengo pertanto che sia giusto dovere ribadire in questa sede che tutti i parlamentari hanno il diritto - se lo ritengono mio avviso anche il dovere di partecipare in maniera attiva al processo di formazione della legge fondamentale del nostro ordinamento legislativo e amministrativo, su cui si regge l’intera impalcatura del funzionamento della pubblica

cioè quella di immaginare che il Parlamento sia un luogo mesto e, se possibile, silenzioso di ratifica delle decisioni che sono già state assunte. In realtà, noi siamo nel luogo della legislazione e la legislazione presuppone il confronto e il confronto presuppone l’iniziativa dei parlamentari, che siano di maggioranza o di opposizione. qualora i parlamentari di maggioranza dovessero trovarsi nella esigenza di dover rappresentare alcune idee, il nostro Gruppo, compatibilmente con le idee che condividiamo dal punto di vista della necessità di modifica, si renderà disponibile a svolgere una funzione a svolgere una funzione di asilo politico per quei parlamentari di destra che vorranno esprimere una loro opinione in materia. La ringrazio e ribadisco quello che ho già detto al suo collega. Io sono sicuro che avranno gradito questa sua opera di difensore dei dei parlamentari, in questo caso dei senatori, di maggioranza, ma nessuno ha mai messo in dubbio la facoltà, ove lo ritenessero, quel che è più importante è che nessuno ha mai neanche ipotizzato di limitare le facoltà

nel convincimento di garantire tutti i senatori di maggioranza e di opposizione nelle loro facoltà concesse dal Regolamento. Nel contempo devo dire che queste preoccupazioni non le ho, perché è di tutta evidenza che qualunque annuncio di tipo politico non può limitare minimamente la libera decisione di ciascun senatore.

di attribuzione III. Discussione del disegno di legge: Deputato MOLINARI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

IV. Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge: